Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione di instabilità politica che caratterizza il Nord Africa e, in particolare, i recenti avvenimenti che hanno interessato la Tunisia e la Libia hanno causato una massiccia ondata di sbarchi sulle coste italiane. Sulle isole di Lampedusa, Linosa e Lampione, dal 1° gennaio al 9 marzo di quest'anno, risultano sbarcati complessivamente 8.104 immigrati di sedicente nazionalità tunisina, di cui 7.869 uomini, 39 donne e 196 minori, a seguito di 125 episodi di sbarco. Sulla sola isola di Lampedusa sono sbarcati 7.989 immigrati. La situazione ha i connotati di una vera e propria emergenza umanitaria che il Governo ha affrontato con soluzioni concrete ed immediate, che necessitano - considerato l'ampio scenario di crisi - di un impegno ormai ineludibile anche da parte dell'Unione europea. Il dispositivo di prima accoglienza che è stato subito predisposto sull'isola di Lampedusa ha consentito che tutti i migranti fossero assistiti e sottoposti a visita medica, con fornitura di vitto, vestiario e generi di uso personale; prestazioni, queste, assicurate non solo nell'immediatezza degli sbarchi, ma anche durante il soggiorno dei migranti ospitati sull'isola presso strutture alberghiere o presso aree messe a disposizione dal Comune, dalla Capitaneria di porto e dalla parrocchia e - in seguito alla sua riapertura - anche presso il centro di soccorso e prima accoglienza, che, a causa del ridotto flusso di immigranti registrato nel 2010, era attivo per la sola manutenzione ordinaria degli impianti e della struttura. Per ampliare ulteriormente la recettività di posti in Sicilia è stata resa operativa anche la struttura tensostatica sita in Rosolini, in Provincia di Siracusa. I migranti sbarcati a Lampedusa, fin dal loro soggiorno sul molo e poi all'interno del centro di accoglienza - come avviene negli altri centri istituiti sul territorio nazionale - sono stati assistiti dagli operatori dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, della Croce rossa italiana e di "Save the children": le quattro agenzie umanitarie *partner* del Ministero dell'interno nell'ambito del progetto «Praesidium», diretto a rafforzare la capacità di accoglienza e di gestione rispetto ai flussi migratori. Le imponenti dimensioni del fenomeno hanno reso necessario garantire continui ponti aerei per il trasferimento dei cittadini tunisini in altri centri ubicati su tutto il territorio nazionale. Sono stati anche organizzati trasferimenti a mezzo nave verso Porto Empedocle, dove è ubicata una tensostruttura con una capienza di 100-130 posti - gestita dalla Protezione civile regionale - anch'essa finalizzata a garantire la prima accoglienza e l'assistenza sociosanitaria agli immigrati. adeguata assistenza è stata assicurata ai minori collocati nelle 21 strutture di accoglienza ubicate nella Provincia di Agrigento ed autorizzate dalla Regione siciliana. Dal 1° gennaio alla data di ieri sono stati complessivamente trasferiti da Lampedusa e Linosa 6.610 clandestini, condotti in aereo o in nave verso Porto Empedocle, nonché presso i centri per immigrati

Alle strutture destinate all'accoglienza e ubicate sul territorio siciliano presto se ne aggiungerà una nuova, individuata nel corso di una riunione tecnico-operativa tenuta al Viminale il 14 febbraio scorso. Si tratta del «*Residence* degli aranci» di Mineo, in Provincia di Catania (già alloggio per i militari della base NATO di Sigonella e ribattezzato «Villaggio della solidarietà»), presso il quale si sono recati nella giornata del 15 febbraio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno. Tale struttura, che dispone di 1.800 unità abitative e può ospitare fino a 7.000 persone, potrà a breve essere destinata all'accoglienza dei rifugiati. Voglio pertanto precisare che il Governo italiano sta gestendo questa emergenza umanitaria con mezzi ed interventi adeguati e con costi assai elevati che, ad oggi, che, ad oggi, sta fronteggiando da solo. Ma la situazione di grave e crescente instabilità politica nell'area nordafricana (che potrebbe ulteriormente aggravarsi e determinare l'apertura di nuove e consistenti rotte migratorie) rende impellente una mobilitazione dell'Unione europea, anche in considerazione dei riflessi che la crisi regionale determina, non solo sulle dinamiche migratorie, ma anche sulla sicurezza interna, con particolare riferimento al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche. Di fronte ad un simile scenario, che non può essere affrontato con un approccio burocratico, il Governo ha richiesto l'intervento - anche economico di 100 milioni di euro - delle istituzioni europee, proponendo azioni concrete da realizzare nell'immediato e nel medio periodo. È di fondamentale importanza l'applicazione del principio del *burden sharing*, ovvero la suddivisione degli oneri e dei pesi relativi alla gestione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei clandestini. È in questo quadro che deve inserirsi il riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore di quegli immigrati che ne hanno diritto. Voglio, infatti, precisare con riferimento allo specifico quesito formulato dall'onorevole interrogante che gli operatori di «Praesidium» e, in particolare, i rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, presenti sull'isola di Lampedusa come negli altri centri di accoglienza, forniscono le informazioni in materia di protezione internazionale e di presentazione della domanda di asilo, informazioni che sono pubblicizzate anche presso le aree comuni dei centri. Il nostro obiettivo, infatti, oltre a quello di fornire un'assistenza adeguata è quello di valutare l'eventuale *status* di rifugiato di questi immigrati, di rimpatriare coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale e di sistemare adeguatamente i rifugiati, come avviene per tutti quelli che hanno chiesto e ottenuto asilo in Italia. Presso i centri di accoglienza nazionali è stata segnalata la presenza di 2.905 tunisini provenienti da Lampedusa. Di essi, 2.835 hanno chiesto la protezione internazionale (1.389 hanno già formalizzato l'istanza mentre 1.446 lo faranno nei prossimi giorni). Per quanto concerne, infine, le clausole di esclusione dal beneficio della protezione internazionale, richiamate dall'onorevole interrogante (che, come è noto, riguardano la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità ovvero reati particolarmente gravi), faccio presente che tali clausole sono espressamente elencate nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di recepimento della direttiva europea 2004/83/CE sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. E su questi delicati aspetti desidero assicurare l'onorevole interrogante che la sussistenza di una causa di esclusione, a cui consegue il rigetto della domanda, è valutata caso per caso, sulla base di tutti gli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura istruttoria,

fosse abbastanza prevedibile. Bastava pensare al pane che in questi Paesi da tempo viene a mancare in maniera consistente, alla carenza di lavoro in questi Paesi, che arriva al 30-40 per cento, alle angherie che il popolo di questi Paesi ha subito negli ultimi tempi e al primo esodo che si è verificato nei primi giorni di quest'anno.

anche con interventi di tipo umanitario, devo dire che si è trovato del tutto impreparato di fronte a questa immigrazione forte che probabilmente non si poteva ritenere così biblica e condivido questa espressione, perché a mio avviso ancora non abbiamo visto niente di quello che dovrebbe arrivare.

la direttiva del 2008, che doveva essere recepita entro il 26 o 24 dicembre 2010 e che prevedeva particolari condizioni per le espulsioni.

può vedere, sono molto modesti. In virtù e nella logica di questa strategia non si è recepita la direttiva europea e ora ci si appella all'Europa. giustamente anche in relazione alla direttiva comunitaria recepita dal Governo Berlusconi nel 2003. Dico subito che l'Unione di Centro sarà vicina al Governo

immigrazione/esodo che arriverà prestissimo in Italia perché - ripeto - ancora non abbiamo visto nulla. Un mese fa un esponente della Lega diceva

Pensiamo ai tagli macroscopici che sono stati effettuati al pacchetto sicurezza, ai continui disagi che gli uomini delle forze dell'ordine subiscono quotidianamente

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna viene posta all'attenzione del Parlamento la questione delle modalità di ridefinizione dei collegi elettorali della Provincia di Perugia. Come è noto, la materia in questione è disciplinata dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come di recente modificato dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Le tabelle dei collegi elettorali provinciali sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentita previamente la Provincia interessata, in numero corrispondente a quello dei consiglieri provinciali da eleggere, variabile in relazione all'entità demografica della Provincia stessa. Le modifiche normative appena citate, che hanno istituzionalizzato la partecipazione degli enti locali nella definizione degli ambiti territoriali dei collegi provinciali, sono il frutto di delicate valutazioni mirate ad armonizzare diversi criteri quali l'omogeneità di struttura geo-economico-sociale, la contiguità territoriale e l'equilibrio demografico. Il Ministero dell'interno, in fase d'istruzione delle proposte, valuta il rispetto dei criteri della contiguità territoriale e dell'equilibrio demografico rimettendosi, per quanto attiene al criterio dell'omogeneità geo-economico-sociale, alle determinazioni degli uffici periferici, unici depositari di fondati elementi di giudizio. Pertanto, dal quadro normativo che ho appena descritto, emerge chiaramente che il Ministero dell'interno, ai fini di una corretta valutazione delle istanze locali, non può prescindere dalla sintesi che di queste viene fatta in ambito territoriale, sia a livello di Provincia che di prefettura. In relazione agli specifici quesiti posti dall'onorevole interrogante, rispondo all'esito degli accertamenti svolti dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e dalla prefettura di Perugia. Quest'ultima ha elaborato una prima bozza di proposta di riassetto dei collegi uninominali, nel rispetto delle istruzioni e dei criteri predisposti dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Preso atto di segnalazioni provenienti anche da alcuni sindaci, ha inoltrato la predetta bozza al presidente della Provincia, così come previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma

che - riunitesi in seduta congiunta e dopo ampia discussione - hanno provveduto, il 25 ottobre 2010, a redigere un documento. Tale documento, il giorno successivo, è stato trasmesso alla prefettura con una nota del presidente della Provincia, nella quale viene esplicitamente asserito che esso «rappresenta l'avviso dell'Ente». La prefettura, dunque, nel prendere atto della definitività del documento ad essa formalmente trasmesso, ha tenuto nel dovuto conto la volontà dell'organo consiliare e, sulla base di tale volontà, ha operato le sue successive valutazioni sulla modifica della proposta, prima di inviarla al Ministero dell'interno. La prefettura ha quindi modificato la proposta iniziale e predisposto una proposta definitiva, trasmessa il successivo 29 ottobre 2010 al dipartimento degli affari interni e territoriali, che è la struttura dell'amministrazione centrale preposta alla promozione e allo sviluppo della Repubblica delle autonomie, attraverso tutti i necessari compiti di raccordo, supporto e collaborazione con le autonomie territoriali. La proposta è stata in seguito oggetto di rilievi da parte della direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, per l'assenza in due collegi del criterio inderogabile della contiguità territoriale. Sulla base di tali rilievi, è stata modificata e ritrasmessa dalla prefettura al Ministero il 27 novembre 2010, dopo alcuni incontri tenuti personalmente dal prefetto di Perugia con i sindaci di Città di Castello e di Gubbio, interessati dall'ulteriore modifica. In ambito provinciale si è quindi riacceso il dibattito su tale documento: in consiglio provinciale si sono manifestati dissensi sul testo di proposta definitiva e il presidente della Provincia è stato invitato dal consiglio a prendere contatto diretto con il Ministero per ottenere ulteriori modificazioni. Voglio poi precisare che la proposta definitiva non solo è stata adottata dalla prefettura dopo aver sentito la Provincia, ma che tale consultazione ha anche portato a una modifica del documento nel senso richiesto dall'ente territoriale, con nota del presidente del 26 ottobre scorso. Infatti, la Provincia chiedeva che l'area cosiddetta del Trasimeno (formula peraltro piuttosto imprecisa), oggi ripartita in quattro collegi, fosse divisa in «meno di quattro collegi». Ebbene, nella proposta prefettizia tale richiesta è stata accolta in quanto i collegi previsti sono tre e non sono possibili ulteriori riduzioni, in quanto foriere di gravi disarticolazioni nelle aree limitrofe. In secondo luogo, è stata accolta anche l'analoga richiesta della Provincia che auspicava una divisione in «meno di quattro collegi» per l'area dell'unione dei Comuni delle «Terre dell'olio e del Sagrantino» (oggi di due collegi). L'area è stata infatti suddivisa in tre collegi provinciali nella proposta in esame. La Provincia formulava, poi, una generica richiesta di «procedere anche ad una serie di spostamenti di carattere minore che non modificano la sostanza della proposta consegnata», richiesta - anche questa - che può dirsi sostanzialmente accolta, dal momento che la proposta della prefettura è stata modificata rispetto alla sua formulazione iniziale, proprio tenendo conto delle richieste della Provincia. La prefettura non ha potuto invece venire incontro all'ulteriore richiesta di superare il criterio della consistenza demografica - anche al di là della sua eccezionale derogabilità fino al 20 per cento in più o in meno - in favore del concorrente criterio dell'«omogeneità territoriale, culturale, storica e sociale». Voglio a questo proposito precisare che il superamento del criterio della consistenza demografica non è nella disponibilità della singola prefettura (essendovi precise istruzioni ministeriali sul punto), mentre l'adozione del criterio alternativo dell'omogeneità non appare supportato da alcuna concreta indicazione, da parte della Provincia, di modalità alternative di aggregazione. Ne è prova il fatto che la Provincia non ha corredato la propria richiesta di una cartografia alternativa a quella fornita dalla prefettura e ciò per la difficoltà di conciliare i criteri ministeriali, le istanze in sede provinciale e le conseguenze a catena sugli altri collegi. Vi è da aggiungere che, mentre i criteri della contiguità territoriale e dell'equilibrio demografico possono essere valutati a livello centrale dal Ministero dell'interno in fase di istruzione delle proposte, sul parametro dell'omogeneità geo-economico-sociale il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno si rimette alle valutazioni degli uffici periferici in quanto solo a livello territoriale possono essere raccolti fondati elementi di giudizio, come d'altronde è avvenuto anche nel caso di specie. Sebbene il fattore numerico non sia l'unico criterio a dover essere considerato, tuttavia non può essere completamente abbandonato, per ragioni sia di ordine pratico che di ordine giuridico. Al momento si sta valutando la proposta definitiva come formulata dalla prefettura di Perugia in tutte le sue implicazioni. L'amministrazione centrale è disponibile ad acquisire ulteriori elementi e valutazioni che il consiglio provinciale o il presidente della Provincia di Perugia vogliano eventualmente far pervenire, purché si tratti di valutazioni imputabili alla volontà dell'ente provinciale espressa nelle debite forme legali. D'altra parte, pur tenendo conto il più possibile degli interessi espressi dall'ente provinciale, il Ministro dell'interno deve privilegiare, nella sua proposta definitiva, funzionale all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, la considerazione dell'interesse pubblico generale e dei parametri adottati sul resto del territorio nazionale. Sicché, ai fini della delicata decisione finale, è necessaria un'attenta ponderazione di tutti i fattori coinvolti, nella quale devono convergere due visioni complementari: quella generale, che fa capo al dipartimento per gli affari interni e territoriali, e quella locale, di cui si rendono interpreti sia la Provincia che la prefettura. Si tratta pertanto di trovare un giusto punto di equilibrio in modo che nella definizione dei collegi vi sia una giusta ed equilibrata rappresentanza di tutte le componenti, salvaguardando le omogeneità territoriali della Provincia, nei limiti del possibile e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

identica a quella già fornita presso la Camera dei deputati all'onorevole Bocci. Nel frattempo, comunque, è intervenuto un chiarimento da parte della Provincia di Perugia a questo proposito, che mi accingo ad esporre, fatta una breve premessa. Questa interrogazione che ho presentato segue un ordine del giorno del Consiglio provinciale di Perugia del 9 novembre 2010 che esprime parere negativo sulla proposta della prefettura di Perugia in merito alla ridefinizione dei collegi elettorali, in quanto disattende le proposte formulate dalle Commissioni consiliari permanenti congiunte il 25 infatti penalizza la rappresentanza di alcune aree della Provincia senza tenere in conto le omogeneità territoriali e le caratteristiche economico-sociali comuni a queste aree, rispondendo solo al criterio del numero degli abitanti.

e quindi, in qualche modo, il criterio numerico di per sé solo può creare disagi che rischiano di penalizzare una corretta rappresentanza in diverse realtà Per questo era stato messo in evidenza che in alcune aree, cui lei ha fatto riferimento, quali l'area del Trasimeno e l'Unione dei Comuni delle Terre dell'olio e del Sagrantino, dovevano essere ridefinite le circoscrizioni tenendo conto proprio di queste caratteristiche caratteristiche che non sono state tenute in considerazione. A questo punto, la Provincia di Perugia, a seguito della vostra risposta alla Camera dei deputati, ha formulato una precisa richiesta, corredata di cartografia, che implica una minima deroga al criterio della consistenza demografica, chiedendo in particolar modo che il Ministero dell'interno possa prevedere nel collegio n. 3 di Castiglion del Lago il Comune di Piegaro, proprio per ristabilire il principio della omogeneità territoriale.

Penso che in questo modo si possa supportare tale proposta, ed in questa sede non faccio altro che sostenere la richiesta avanzata dalla Provincia.

del bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e l'esigenza - parimenti rilevante a livello costituzionale - della tutela dell'ordine pubblico. L'atto di sindacato ispettivo si incentra sulla manifestazione che avrebbe dovuto tenersi il 28 dicembre 2010 a Civitavecchia, con la partecipazione di circa 200 aderenti al Movimento pastori sardi, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche proprie del loro settore economico. Gli interroganti asseriscono che le forze di polizia avrebbero impedito ai manifestanti di recarsi a Roma - ove era loro intenzione dar luogo ad una manifestazione pacifica davanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - trattenendoli, con un blocco preventivo, nel porto di Civitavecchia, prima del reimbarco, in serata, per Olbia. Si lamenta quindi la violazione dei principi di libera manifestazione del pensiero e di libera circolazione delle persone, stigmatizzata anche dal Consiglio regionale della Sardegna. Prima di ricostruire i fatti voglio subito assicurare agli interroganti che non vi è stata alcuna violazione dei principi costituzionali da parte delle forze di polizia che, anzi, hanno garantito il pieno rispetto dei dettato costituzionale ed hanno applicato la normativa vigente, sia deferendo all'autorità giudiziaria quanti tra i manifestanti si erano resi autori di fatti perseguibili penalmente, sia impedendo il realizzarsi di ulteriori illegalità. L'articolo 17 della Costituzione prevede, infatti, che i promotori di una manifestazione in luogo pubblico hanno l'obbligo di darne preavviso alle autorità, le quali possono vietarla per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La Carta costituzionale si preoccupa, pertanto, di operare un bilanciamento tra il diritto di riunione - che il primo comma dell'articolo 17 esige sia sempre esercitato in modo pacifico e senza armi e la necessità di garantire che tali riunioni non mettano a rischio altri fondamentali diritti costituzionali, quali appunto la sicurezza e l'incolumità pubblica. Proprio a tale scopo, il Costituente il preavviso alle autorità di pubblica sicurezza, cui compete valutare, in base all'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le circostanze e le condizioni che, nel caso concreto, appaiono necessarie per consentire riunioni e manifestazioni oppure, al contrario, vietarle o consentirne lo svolgimento secondo modalità diverse da quelle previste dagli organizzatori. Dagli accertamenti esperiti attraverso gli uffici competenti è emerso che la manifestazione dei pastori sardi non è stata in alcun modo preavvisata alle competenti autorità. Anzi, in più momenti della giornata del 28 dicembre, i manifestanti hanno tentato di dare vita ad una pluralità di manifestazioni non preavvisate. Ritengo ora necessaria una dettagliata ricostruzione dei fatti. Il 27 novembre 2010 la DIGOS della questura di Roma riceveva la notizia che aderenti al Movimento pastori sardi avevano intenzione di raggiungere la Capitale per richiamare l'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa - in maniera eclatante - sulla crisi della pastorizia sarda. La notizia è stata poi confermata dalla questura di Cagliari, secondo cui numerosi aderenti avrebbero raggiunto Civitavecchia con la motonave Tirrenia, guidati dal loro leader, il signor Felice Floris. infatti, alle 5,45 del successivo 28 dicembre, circa 200 pastori giungevano a Civitavecchia con la motonave Tirrenia e, appena scesi, dopo essersi compattati, sventolando bandiere, davano luogo, già all'interno del porto, ad una prima manifestazione non preavvisata. Il funzionario della Polizia di Stato al quale, alla luce delle informazioni previamente raccolte, era stato affidato il compito di predisporre un adeguato servizio di ordine e sicurezza pubblica, prendeva subito contatto con il signor Floris. Quest'ultimo, nella qualità di portavoce del Movimento, esplicitava l'intenzione di raggiungere Roma con cinque pullman in arrivo al porto e di effettuare inoltre un blocco stradale sul grande raccordo anulare, all'altezza della Bufalotta, ove li avrebbe attesi la stampa. Una serie di elementi facevano apparire del tutto verosimili tali intenzioni: innanzitutto, effettivamente cinque pullman si trovavano in attesa di prelevare i dimostranti; inoltre, in precedenza, sia il signor Floris sia un'altra portavoce del Movimento avevano preannunciato eclatanti azioni dimostrative a Roma e Bruxelles. risultavano confermate *ex post* dal rinvenimento presso il porto di Civitavecchia di numerosi volantini indirizzati agli automobilisti romani, con cui i manifestanti chiedevano scusa per il disagio arrecato con il blocco stradale. Sebbene avvisati che il blocco stradale non sarebbe stato consentito in quanto penalmente rilevante, i dimostranti, per tutta risposta, bloccavano per circa un'ora lo sbarco degli automezzi dalla motonave Tirrenia. A questo punto, il personale della Polizia di Stato tentava di venire incontro alle esigenze dei dimostranti, prospettando loro la possibilità di autorizzare una manifestazione a Civitavecchia, a condizione che fosse presentato un regolare preavviso. I manifestanti opponevano un netto rifiuto, ribadendo l'intenzione di raggiungere ad ogni costo Roma ed anzi preannunciando la volontà di bloccare la vicina via Aurelia. Veniva quindi effettuato uno schieramento di forza pubblica, per evitare la dispersione dei manifestanti, consentire alla polizia scientifica di effettuare dei filmati e procedere quindi alla formale identificazione dei manifestanti stessi. Invitati a fornire le generalità, i dimostranti si rifiutavano, tentando anzi con la violenza di forzare il cordone della forza pubblica e facendo cadere a terra alcuni poliziotti. In questa fase di concitazione, veniva bloccato il leader del gruppo che, dopo l'identificazione ed attesa la decisione di procedere nei loro confronti in stato di libertà, veniva immediatamente rilasciato. A questo punto i manifestanti si disperdevano, radunandosi in piccoli gruppi nell'area portuale e raggiungendo i servizi, i bar o, alcuni, i pullman che li attendevano. Proprio in questa fase si apprendeva l'intenzione dei manifestanti di raggiungere la stazione ferroviaria di Civitavecchia, dove dapprima, verso le ore 9, erano giunte nove persone, tutte identificate. Dopo qualche minuto, giungeva una trentina di dimostranti, i quali, esibendo i fazzoletti del Movimento e agitando bandiere, stavano già effettuando un'ulteriore manifestazione non preavvisata, in parte marciando sulla sede stradale. Le forze di polizia presenti sul posto non consentivano la prosecuzione dell'iniziativa, dal momento che appariva evidente l'intenzione dei manifestanti di raggiungere la Capitale per attuare la preannunciata manifestazione. I dimostranti venivano invitati a tornare insieme al resto del gruppo presso l'area portuale, invito cui hanno aderito pur mostrando disappunto. Nella serata, tutti i manifestanti si sono imbarcati alla volta di Olbia. Il signor Floris è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di manifestazione non preavvisata. Sono inoltre in corso indagini per risalire, tramite le riprese della polizia scientifica, ai responsabili delle illegalità commesse durante i disordini. Tutto ciò premesso, voglio ribadire che la gestione del servizio di ordine pubblico è stata condotta con prudenza ed equilibrio, secondo un modulo operativo già sperimentato con successo, che mira a contenere le tensioni evitandone di più gravi. A titolo esemplificativo, voglio richiamare alcune scelte operate dalle forze di polizia durante la giornata del 28 dicembre, volte ad attenuare il più possibile la conflittualità, quali la proposta - fatta ai dimostranti e da questi rifiutata - di tenere una manifestazione a Civitavecchia; la decisione di non identificare tutti i manifestanti; i ripetuti tentativi di interloquire con i portavoce del Movimento e di spiegare il disvalore penale delle azioni programmate. Voglio infine assicurare agli interroganti che le autorità di pubblica sicurezza, in questa come in altre circostanze, svolgono con attenzione il delicato compito di garantire a tutti i cittadini il pacifico esplicarsi del diritto di riunione e di libera manifestazione del pensiero. In nome di tali diritti, non è ammissibile giustificare la violazione di altri che la stessa Costituzione ha posto come limiti non valicabili, né, tanto meno, avallare comportamenti che l'ordinamento ha già valutato come penalmente rilevanti, in quanto pericolosi per l'ordinata convivenza civile e la sicurezza pubblica, quali il reato di manifestazione non preavvisata o di Signor Sottosegretario, se dovessi dirle che lei ha assolto sforzandosi di sfuggire alla patina di insopportabile sapore burocratico che c'è nelle risposte alle interrogazioni, e che quindi sono soddisfatto della sua risposta, le direi una grandissima bugia, ma non sono capace di farlo.

come i *farmers* americani di Steinbeck, il loro "Furore", ma potrebbe anche raccontare la disperazione che li porta a saltare un mare,

Costoro, quelli che sono arrivati a Civitavecchia, dovevano raccontare, anche per conto di chi era rimasto a lavorare, lo stato di disperazione delle campagne sarde. Queste persone lavorano vendendo un prodotto che viene loro acquistato dall'industria a 65 centesimi al litro: il latte delle pecore. Governo sono più interessate ad altre produzioni lattiere, ma il latte di pecora vale 65 centesimi al litro, meno della metà di un litro di benzina. diverse migliaia di aziende in questo momento in Sardegna sono all'asta. Non le aziende frutto dell'arricchimento di un fortunato ciclo economico ma quelle ereditate dai padri, ereditate dai padri, che magari sono andati sventolando le stesse bandiere, forse quella con i quattro mori cui lei ha fatto riferimento nel suo discorso, nel suo discorso, per fare questo Paese unito in tutto il ciclo delle guerre che hanno portato alla sua Unità e che quest'anno, tra qualche giorno, celebreremo Quindi, mi consenta di dirlo con parole che non sono mie, bisogna considerare veramente "il mare come la fine del mondo per capire quello che è successo" e "aver sentito pronunciare il nome di Roma come quello di un luogo onnipotente e lontanissimo", dove si risolvono i problemi: questo volevano quei 200 signori e signore, ragazzi e ragazze, che, svegliatisi presto, hanno preso il traghetto e fatto le loro 12-14 ore di nave arrivando a Civitavecchia. Volevano venire a dare dei volantini a Roma davanti alla sede del loro Governo, non del Governo di un Paese ospite e straniero. Presidente Nania, lei ha detto, annunciando l'interrogazione, che essa riguardava una manifestazione di "pastori sardi": pastori italiani, poi certo pastori sardi. Vede, la lettura che lei dà, signor Sottosegretario, del del modo con cui si devono bilanciare i valori costituzionali del diritto di manifestare la propria critica

fondamentale che questa interrogazione, firmata da tutti i senatori della Sardegna, di centrodestra e centrosinistra, ha voluto mettere in rilievo. di tensione probabilmente si risolvono meglio (visto anche che il problema di ordine pubblico era dato da 200 persone, non da 200.000, perché se non diamo questo dato probabilmente capiamo

questa Roma importante, onnipotente, eterna, grande che risolve i problemi. Invece no, non li si è nemmeno voluti ascoltare.